Fabrizio Palenzona, vicepresidente di Unicredit, che ha affari anche nel settore delle autostrade, essendo presidente di Aiscat, la concessionaria che riunisce tutti i i gestori autostradali. Gli aeroporti di Roma non brillano per efficienza. I sondaggi svolti

per cui i profitti sono privati e gli oneri sono pubblici, questa volta a carico dei passeggeri. Noi siamo rimasti molto stupiti da questo aumento di 3 euro

un monitoraggio e un controllo sulla puntualità. Tra l'altro, l'ultima inchiesta pubblicata il 10 marzo scorso dal settimanale «L'Espresso» conferma questa situazione di disagio si stigmatizza l'inidoneità del servizio di acquisizione e consegna dei bagagli dei viaggiatori e si riportano episodi incompatibili con l'attenzione che dovrebbe essere riservata alla gestione di tale aspetto all'interno del principale aeroporto della capitale.

(Madrid-Barcellona ha 32.418 voli all'anno, Fiumicino-Linate è seconda con 21.507)

questi "capitani coraggiosi" che - ripeto - sono adusi a privatizzare i profitti e a socializzare le perdite. Ci auguriamo che vengano effettuati i controlli, che ci sia un attento monitoraggio

i disservizi registrati presso l'aeroporto di Fiumicino nell'anno 2009 e l'anticipazione tariffaria dei diritti aeroportuali per l'imbarco passeggeri, così come stabilito dalla legge finanziaria 2010. In riferimento alla prima tematica, si rappresenta che l'anno 2009 è stato caratterizzato da difficoltà dovute al particolare momento congiunturale connesso alla nota vicenda Alitalia. Per far fronte a detta situazione, sono state indette una serie di riunioni con i soggetti interessati e sono stati effettuati *audit* di verifica. Nel mese di novembre si sono tenuti gli *audit* conclusivi nei confronti degli *handler* e del gestore stesso, nel corso dei quali è stato riscontrato il rientro dalle criticità precedentemente emerse. Dalle verifiche effettuate dall'ENAC, infatti, è emersa una situazione di sensibile miglioramento rispetto al periodo estivo. Tale *trend* di miglioramento è confermato anche dai recenti dati registrati nei primi mesi del 2010 relativamente ai disservizi riguardanti la gestione dei bagagli. Ciò grazie alle azioni infrastrutturali poste in essere dai gestori aeroportuali e da Alitalia stessa presso lo scalo romano. Pertanto, allo stato attuale non si registrano situazioni negative, se non quelle tipiche di uno scalo internazionale di grandi dimensioni come quello di Fiumicino. In riferimento quindi alle tariffe aeroportuali, occorre fare alcune considerazioni preliminari. Nelle more dell'applicazione della direttiva 2009/12/CE e nelle more della stipula dei contratti di programma di cui al paragrafo 5.2 della delibera CIPE n. 38 del 2007 ed all'articolo 17, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, la legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010) ha autorizzato, a decorrere dall'anno 2010, un'anticipazione tariffaria dei diritti aeroportuali per l'imbarco passeggeri nel limite massimo di 3 euro. Come noto, si è intervenuti con tale disposizione al fine di accelerare la realizzazione di investimenti infrastrutturali da parte dei gestori aeroportuali, prevedendo al contempo che la misura così determinata resterà in vigore sino alla stipula dei contratti di programma determinando, in tal modo, il carattere transitorio della disposizione stessa. L'obiettivo, quindi, di tale disposizione è quello di consentire alle società di gestione aeroportuale, pur in una fase di stallo congiunturale e di stagnazione del traffico, di avviare la realizzazione di quegli interventi necessari all'ammodernamento delle infrastrutture aeroportuali ed il loro adeguamento ai requisiti di sicurezza operativa prescritti dalle vigenti normative o al mantenimento della certificazione aeroportuale, nonché al recupero dei livelli di servizio offerti all'utenza. Va in merito precisato che l'anticipazione accordata dalla legge finanziaria 2010 non è stabilita in una quota fissa di 3 euro bensì non può superare il limite massimo di 3 euro a passeggero in partenza dallo scalo interessato. Tale disposizione, in linea con il principio di "non discriminazione" previsto all'articolo 3 della direttiva 2009/12/CE, si applica a tutte le società affidatarie della gestione aeroportuale, anche a titolo parziale precario, che presentino istanza di ammissione all'ENAC corredata da un piano di sviluppo e ammodernamento aeroportuale con allegato elenco delle opere ritenute urgenti ed indifferibili nonché del relativo cronoprogramma. di accedere a modalità di pre-finanziamento degli investimenti infrastrutturali urgenti relativi all'esercizio delle attività aeronautiche, attraverso l'aumento massimo di 3 euro per passeggero in partenza in voli all'interno ed all'esterno del territorio dell'Unione europea. Va tuttavia ricordato che l'ammissione all'anticipazione tariffaria è condizionata alla validazione tecnica da parte dell'ENAC degli interventi programmati - in ordine alla loro cantierabilità, necessità, urgenza, congruità e sostenibilità economica ed è rapportata al costo delle opere. Sulla base dell'intervenuta validazione tecnica, l'ENAC propone quindi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'economia l'entità della «anticipazione tariffaria» annuale da accordare, previo parere favorevole del CIPE-NARS, alla singola società di gestione. Le entrate riscosse per effetto di tale procedura devono essere accantonate dalla società concessionaria in apposito fondo vincolato iscritto nello stato patrimoniale fintanto che, a seguito del vaglio dell'ENAC sullo stato degli adempimenti connessi alle lavorazioni programmate ed eseguite (SAL), ne sarà autorizzato lo svincolo. Lo svincolo delle somme accantonate viene pertanto accordato a fronte dell'effettiva realizzazione da parte delle società concessionarie degli interventi urgenti ammessi e nei limiti dei SAL convalidati dall'ENAC. È opportuno rilevare che il meccanismo dell'anticipazione tariffaria prevede dei casi di decadenza della stessa della stessa a seguito della mancata presentazione da parte della società concessionaria, nel termine di sei mesi dalla data di validazione tecnica da parte dell'ENAC, dei piani quadriennali di sviluppo, di tutta la documentazione necessaria alla stipula dei contratti di programma. Un'altra causa di decadenza è derivata dalla mancata stipula del contratto di programma entro i 18 mesi decorrenti dalla data di validazione tecnica da parte dell'ENAC del piano quadriennale nonché dal mancato avvio della realizzazione delle opere nei termini e nelle modalità fissate dal piano di sviluppo e dal relativo cronoprogramma. Alla luce di quanto illustrato, l'anticipazione tariffaria costituisce un «provvedimento ponte» che si propone di attivare da parte dei gestori aeroportuali un flusso di investimenti in attesa della stipula dei contratti di programma tra ENAC e le singole società di gestione aeroportuale. In ultima analisi, preme rilevare che, trattandosi di provvedimento temporaneo, pochi gestori hanno ad oggi presentato istanza in tal senso.

Prendiamo atto che vi sarebbe stato un lieve miglioramento della qualità dei servizi offerti da questo importante scalo non solo della capitale ma dell'intero tuttavia, non possiamo ritenerci soddisfatti per una semplice ragione. I capitalisti si chiamano così in tutti i Paesi del mondo, perché sono coloro che tirano fuori dalle loro tasche i cosiddetti capitali di rischio; li tirano fuori per intraprendere la loro attività,

Passo a rispondere congiuntamente agli atti ispettivi dei senatori Nerozzi e Carlino, inerenti le vicende occupazionali dei dipendenti dell'ex gruppo Compagnia italiana turismo

il commissario straordinario del gruppo CIT è stato autorizzato, all'esito della procedura ad evidenza pubblica di cessione dell'intero complesso aziendale, ad accettare l'offerta di acquisto presentata da Soglia Hotel Group s.r.l. La stipula del contratto di cessione è avvenuta in due soluzioni. Dapprima, infatti, sono stati ceduti a Soglia Hotel Group s.r.l. la componente mobiliare del patrimonio ed il personale impiegato presso la CIT; successivamente, si è provveduto alla cessione del patrimonio immobiliare alla società Sistema Vacanze s.p.a.,

la cessione del 90 per cento del capitale di Sistema Vacanze alla società Morera s.r.l., nonché il mancato pagamento, per diversi mesi, degli stipendi ai propri dipendenti. Conseguentemente, il commissario ha esperito azione legale nei confronti del gruppo Soglia e di Sistema Vacanze s.p.a., finalizzata all'accertamento delle inadempienze contrattuali ed al conseguente pagamento delle penali previste. Al riguardo, sono in grado di informare che la quasi totalità delle retribuzioni spettanti al personale sono state corrisposte, residuando invece importi sul pagamento del TFR. Tanto premesso, faccio presente che la Soglia Hotel Group s.r.l. ha beneficiato per l'intera annualità del 2009 del trattamento di CIGS per crisi aziendale per complessive 270 unità. Informo inoltre che lo scorso 26 gennaio è stata avviata la procedura per la concessione del trattamento di CIG in deroga alla normativa vigente, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2010, nei confronti dell'intero organico della Soglia Hotel Group (pari a 269 unità). Al riguardo, faccio presente che il decreto di ammissione al trattamento, da me sottoscritto, è stato trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze per la controfirma. In conclusione, nell'informare, sulla base di quanto comunicato dal competente Ministero dello sviluppo economico, che lo scorso 2 febbraio il gruppo Soglia è stato posto in liquidazione, non posso che confermare la più ampia disponibilità a valutare, qualora richiesto, ogni possibile, ulteriore iniziativa diretta a tutelare la posizione dei lavoratori e delle loro famiglie.

In gennaio di quest'anno sia Soglia Group che i sindacati hanno sollecitato un incontro presso il Ministero dello sviluppo economico ed un intervento da parte di quest'ultimo con la Sistema Vacanze s.p.a. Soglia Group sollecitava la salvaguardia delle realtà aziendali ex CIT e stigmatizzava il comportamento di Sistema Vacanze e delle di lei controllanti, le quali, ad oggi, non hanno fornito alcun riscontro, nonostante la rilevantissima importanza della questione, che mette in serio pericolo il posto di lavoro di oltre 250 persone. Sono lavoratori che hanno vissuto nell'incertezza della cassa integrazione e nella speranza di una ripresa del lavoro, almeno attraverso i villaggi ex Vacanze Italiane (ex CIT), passati di mano in mano attraverso accordi tra vecchie e nuove società, oggi affidati in gestione alla società Mondotondo. Villaggi nati tra le contestazioni, cresciuti tra i debiti, venduti e rivenduti, localizzati soprattutto al Sud, in Puglia e in Sicilia, Regioni dove il rilancio del turismo potrebbe fare molto sia all'economia sia al tasso di occupazione. Invece, in questi villaggi, in particolare in quello di Scanzano Jonico, siamo davanti ad un nuovo capitolo nero per i lavoratori. notizia è di questi giorni - le maestranze dei villaggi hanno manifestato in quanto sembrerebbe che il nuovo gestore (Mondotondo) intenda assumere il personale stagionale con modi al limite della regolarità, utilizzando lavoratori anche di cooperative non del territorio.

testimonianze di lavoratrici a cui è stato proposto lavoro *part-time* attraverso una cooperativa, in parte pagato in nero. Signor Sottosegretario, fermo restando che gran parte degli interventi avrebbero dovuto essere messi in atto prima,

ringrazio il sottosegretario Viespoli per la sua attenzione ai problemi delle crisi aziendale e per aver prevenuto

i problemi, cosa che si fa insieme. Il Governo ovviamente poi ne trae beneficio, come chi sostiene le cause, in questo caso, di questi lavoratori. Quindi, un'attenzione maggiore e un modo di lavorare che renda meno inutile il lavoro di noi tutti, io credo sarebbero opportuni. Nel merito solo due considerazioni. Queste crisi aziendali che non coinvolgono un grandissimo numero di addetti, ma che pure riguardano centinaia di addetti, e quindi di famiglie,

assai complicati. La senatrice Carlino mi ha preceduto su alcune considerazioni: bisogna seguire tutto l'*iter* della ex CIT e di questi lavoratori, perché il rischio è di trovarci di fronte ad aziende a diversi passaggi, magari ricevono soldi pubblici e poi i lavoratori che dovrebbero beneficiare di ciò non ne beneficiano,